Il relatore, senatore Ostellari, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi

ampiamente noto - torna nuovamente all'esame di quest'Assemblea. Il testo è stato modificato dalla Camera limitatamente ai profili di copertura finanziaria. Il provvedimento consta di nove articoli,

La previsione estende le norme sul gratuito patrocinio, sui criteri e sulle modalità di liquidazione, e quindi dei compensi e delle spese per la difesa, a favore della persona nei cui confronti siano stati disposti l'archiviazione, il proscioglimento o il non luogo a procedere per i fatti commessi in condizioni di legittima difesa o eccesso colposo. Proprio la norma di copertura è stata oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati: rispetto al testo approvato dal Senato nell'ottobre dell'anno scorso, che prevedeva una copertura anche per quell'esercizio finanziario, l'altro ramo del Parlamento è intervenuto facendo decorrere l'onere ovviamente dal 2019 e adeguando, di conseguenza, la copertura finanziaria al corrente triennio 2019-2021. Tale modifica è stata resa necessaria in quanto, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, le quote dei fondi speciali di parte corrente riferita a provvedimenti non approvati in via definitiva entro la fine dell'anno costituiscono economia di bilancio. Questo è il contenuto tecnico della riforma che andiamo a esaminare oggi, per quanto riguarda l'articolo 8. Prima dell'ultimo atto, nel quale il percorso si concluderà, concedetemi una precisazione sul concetto sul concetto di difesa, che non è offesa, ma il suo contrario: sembra banale, eppure in pochi, commentando questa riforma, hanno compreso la differenza ontologica che sussiste tra difendere, difendersi e offendere. Se qualcuno si introduce nel mio domicilio senza il mio consenso, sta già minacciando la mia vita e mettendo a repentaglio quella dei miei cari, perché ha scelto di oltrepassare un limite, un limite, commettendo un'azione che ha suscitato in me il fondato sospetto che non si fermerà di fronte a nulla, anche a rischio di pregiudicare la mia incolumità e quella di chi mi sta vicino. a casa mia con violenza e senza chiedere permesso, non solo mi ha messo nelle condizioni di scansarmi, scappare o valutare il suo grado di pericolosità, posto che io ci riesca, ma ha fatto molto di più: mi ha necessariamente posto nella condizione,

Quale dovrebbe essere, allora, la posizione dello Stato di fronte a ciò? Per qualcuno dovrebbe essere anzitutto di dubbio, incertezza e sospetto; per noi no: noi no: la difesa, in queste circostanze e in questi luoghi, dev'essere sempre considerata, salvo prova contraria, pienamente legittima. Se mi difendo, la giurisdizione dello Stato non viene meno, anzi, rimane proprio per evitare l'abuso del diritto e anche da domani allo Stato spetta e spetterà il compito di valutare se l'esercizio della difesa non diventi una scusa per realizzare un'offesa immotivata. Cari colleghi, quante volte abbiamo sentito dire che con questa riforma vogliamo sostituire l'individuo allo Stato? Tante, troppe volte. Lo dico chiaramente: da domani il domicilio privato degli italiani non diventerà il *far west*; non sarà un ambito dove vale tutto; non si trasformerà in uno spazio estraneo al diritto; sarà invece un territorio in cui - come in tutti gli altri dell'agire umano la legge distingue con chiarezza chi è la vittima e chi è il carnefice, chi è nel giusto e chi non lo è e dove i magistrati realizzano e continueranno a realizzare la giurisdizione dello Stato, con una differenza rispetto al passato: in situazioni ben definite, il cittadino che si difende da un'offesa commette sempre un'azione legittima. Reagire a una minaccia concreta per eliminare un pericolo, nelle forme della mia spontaneità, in situazioni e stati d'animo che non ho scelto né cagionato, non può essere una colpa, ma è un diritto e, forse, anche un dovere. Cari colleghi, il testo che siamo chiamati a votare ha quindi subìto solo quell'unica modifica di cui abbiamo detto prima. Si tratta di un testo che ha unificato numerosi disegni di legge e accolto diverse sollecitazioni giunte in Commissione da parte sia di coloro che intendiamo tutelare - mi riferisco ai cittadini perbene, che sono stati costretti a difendersi sia dei rappresentanti di associazioni, magistrati e avvocati. È un testo su cui si è lavorato con scrupolo e coscienza,

riforma - se oggi abbiamo di fronte un testo di buon senso, una riforma attesa ed equilibrata. Quindi, cari colleghi, andiamo ad approvarla.

*(FdI)*. Signor Presidente, signori del Governo, cari colleghi, ho ascoltato attentamente le parole del relatore e le condivido pienamente. Peccato che alle parole del relatore faccia seguito un testo legislativo che presenta ancora - a nostro avviso - parecchie lacune.

che, nel caso di eccesso colposo, limita il risarcimento a un'equa indennità lasciata all'equo apprezzamento del giudice. Peccato - ma questo non dipende dal legislatore - che questa riforma valga solo per il futuro, non trattandosi di norma penale più favorevole. sarebbe servito più coraggio, caro relatore, ad esempio ascoltando di più le proposte che da più parti sono venute - soprattutto da Fratelli d'Italia - in ordine ad alcune semplici considerazioni che vado brevemente a esemplificare.

con la norma che stiamo per approvare. Se i due anziani coniugi aggrediti e seviziati in casa loro si fossero difesi con un'arma di tal genere, sarebbero stati condannati per omicidio e, in base alla norma che questa maggioranza ha approvato, non solo sarebbero stati tenuti a risarcire il danno, ma addirittura gli aggressori, una volta usciti dal carcere, avrebbero il reddito di cittadinanza. Abbiamo presentato un emendamento per risolvere questa chiara incongruenza ed andiamo avanti. L'articolo 52, al comma 2, è rimasto inalterato, tranne che per l'aggiunta di quel «sempre» che non occorre un giurista per capire che non ha alcuna portata normativa. Ebbene, in base a questo comma 2, chi usa l'arma per difendere la propria incolumità è assistito dalla proporzione tra la difesa e l'offesa; chi invece usa l'arma per difendere i beni propri o altrui non è assistito da tale presunzione, ma deve dimostrare in primo luogo che non vi è stata desistenza da parte dell'aggressore e, in secondo luogo, che vi era pericolo di aggressione. Ma io vi chiedo come fa chi viene aggredito in casa propria a sapere se chi entra con la violenza vuole aggredirlo personalmente o vuole semplicemente rubargli l'argenteria:

quando l'aggredito avrà accertato se le intenzioni erano queste, sarà già morto. Abbiamo presentato un emendamento per risolvere questa incongruenza ed un altro esempio: all'articolo 55 il nuovo comma introdotto prevede che, nei casi di cui alla difesa domiciliare, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto della salvaguardia della propria o altrui incolumità, e non vi è alcun riferimento ai beni proprio o altrui di cui all'articolo 52. E allora torniamo da capo: come fa una persona che sta in casa e subisce l'intrusione a sapere se è in pericolo la sua incolumità o se sono in pericolo soltanto i suoi beni? Quando lo capisce, è già morto. E ancora, sempre all'articolo 55 si dice che la punibilità è esclusa se chi si difende è in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo. Ma chi stabilisce il grave turbamento? Tutti capiscono che si lascia un'enorme discrezionalità al giudice. Lasciare un'enorme discrezionalità al giudice vuol dire che anche in futuro coloro che purtroppo saranno costretti a difendersi dovranno subire ancora una volta il penoso calvario giudiziario che invece questa legge si propone di evitargli. Fratelli d'Italia aveva proposto di far riferimento, per escludere la punibilità, non allo stato soggettivo dell'aggredito, che - tutti lo capiscono - per sua stessa natura è molto opinabile

criterio certamente più oggettivo e più facilmente dimostrabile. Anche questo emendamento è stato respinto, come quello che voleva includere - come ho detto prima - anche la salvaguardia dei propri beni e non soltanto della propria incolumità. Ancora: nella legge che noi, comunque, oggi approviamo rimane il riferimento alla necessità della difesa e rimane il riferimento all'attualità del pericolo. Ebbene, cosa dice la giurisprudenza? Dice che, a prescindere dal fatto che noi dichiariamo che la proporzione tra offesa e difesa è sempre presunta, il giudice, quando vuole valutare la necessità della difesa, deve necessariamente fare riferimento sia al rapporto tra i diversi beni sacrificabili - quello dell'aggredito e quello dell'aggressore - sia al rapporto tra gli strumenti di difesa e di offesa a disposizione delle due parti opposte. risultato è che, anche in questo caso, si lascia un'amplissima discrezionalità al giudice. Anche in questo caso, il calvario giudiziario sarà tutt'altro che evitato. Occorreva affermare - secondo noi - signor Presidente, colleghi, che la difesa domiciliare è sempre un diritto. Bisognava avere questo coraggio. Ma gli amici della Lega non hanno avuto questo coraggio. Fino a ieri avrei fatto un appello ai colleghi della Lega a ragionare su queste circostanze. Dopo che ieri, però, i colleghi della Lega hanno votato la concessione del reddito di cittadinanza anche ai delinquenti, ai malfattori e ai criminali, mi sono convinto che ormai non c'è più differenza, in questa maggioranza, tra 5 Stelle. E mi sono convinto che, purtroppo, la strada per affermare davvero che la difesa è un diritto è ancora molto lunga.

Noi vogliamo mettere in evidenza semplicemente due questioni di fondo. La prima questione riguarda il fatto che è vero che è stata fatta molta confusione - su questo

Questa è una buona legge, sicuramente migliorabile - come ha detto il senatore Balboni - e lo è perché è di natura parlamentare. Essa è venuta fuori, cioè, dalla sintesi di varie proposte di legge, sia leghiste, di Forza Italia e ed è stata elaborata lungamente in Commissione, con una serie di audizioni, che hanno portato a un testo normativo di natura parlamentare. Credo che esso sia ben approfondito e per questo lo voglio rimarcare. Anche «il manifesto», qualche giorno fa, riportava che ci sarebbe stata una specie di festa in pompa magna del Ministro dell'interno. Io credo che qui si tratti non di festeggiare nulla, ma di dare atto del fatto che, quando il Parlamento è messo nelle condizioni

noi stiamo per votare un testo dove sono stati stabiliti alcuni princìpi, vale a dire che esiste sempre una proporzione tra la difesa e l'offesa

dove si pensa che magari ci si compra una pistola e si risolvono tutti i problemi; noi siamo un Paese, permettetemi di dirlo, di gente perbene, cioè di persone che vogliono semplicemente lavorare in pace nel proprio negozio e stare in pace nella propria casa. vogliono che lo Stato faccia il proprio mestiere e considerano quindi la legittima difesa e la relativa previsione normativa come la *ratio* estrema nei casi peggiori che possono capitare.

quindi che va bene questa legge, ma è un primo passo, un passo fatto bene per i motivi che dicevo prima, perché di natura parlamentare, ma c'è ancora tantissimo lavoro da fare.

la primogenitura, ma la sostanza del provvedimento che oggi andiamo ad approvare, una sostanza che ha un quadro normativo di riferimento preciso, l'istituto della legittima difesa, *ex* articolo 52 del codice penale, collocato tra le cause di giustificazione del reato e fondato sulla necessità di autotutela della persona nel momento di un'assenza della tutela ordinaria.

«proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa». Qui entra in gioco l'aspetto controverso e delicato della proporzionalità, ovvero della sussistenza di un rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa cui fa riferimento l'articolo 614

quello che è stato scritto e scolpito nel contratto di Governo Grillo-leghista e che cito testualmente, perché ci serve per fare memoria. Si legge: «In considerazione del principio dell'inviolabilità della proprietà privata, si prevede la riforma ed estensione della legittima difesa domiciliare eliminando gli elementi di incertezza interpretativa (con riferimento in particolare alla valutazione della proporzionalità tra difesa e offesa) che pregiudicano la piena tutela della persona che ha subìto intrusione nella propria abitazione e nel proprio luogo di lavoro». Qual è, però, il punto? È proprio il contratto Grillo-leghista al quale ho fatto necessariamente riferimento: noi infatti abbiamo seguito il provvedimento in Commissione giustizia, sia qui in Senato che alla Camera, e avremmo voluto

Noi riteniamo che di questo confronto dialettico la materia più sensibile del provvedimento ne abbia risentito in peggio. Naturalmente vale quanto è stato già detto dal mio collega Balboni, ma voglio sottolinearlo, perché chi è costretto a difendersi ora sarà più tutelato (questo è evidente), chi è vittima di un'aggressione sarà più tutelato e soprattutto verranno risparmiati alle vittime anni e anni di calvario giudiziario, di spese legali e di spese di risarcimento ai parenti del rapinatore. in Aula oggi sono stati invitati alcuni esponenti delle associazioni delle vittime, cioè di coloro che hanno subìto o ancora stanno subendo calvari giudiziari per eccesso colposo di legittima difesa. evidentemente - come è già stato notato - resta inevitabile l'apertura di un'inchiesta giudiziaria a carico di chi si difende in casa propria. Al di là del perimetro strettamente legislativo, le maglie sono allora più strette, è vero e ne siamo contenti; infatti voteremo in modo favorevole questo provvedimento. Ma resta ampia ampia ed eccessiva la discrezionalità del giudice nella valutazione della proporzionalità tra offesa e difesa. Quando sento parlare - lo ha detto anche il mio collega Balboni - di quello che resta di quello stato soggettivo, non può non venirmi in mente e nel cuore quello di incredibile che alcune sentenze, anche ultimamente, ci hanno restituito, parlando di tempeste emotive nei casi di femminicidio, dando a questa evidenza una prova dei fatti e trasformando lo stato emotivo di tempesta in una attenuante. *(Applausi dai

vulnerabilità in quei margini di discrezionalità nella valutazione della proporzionalità. Siamo sicuri che la sostanza cambi? Siamo sicuri che stiamo consegnando uno strumento legislativo che poi non veda comunque chi ha subìto un'aggressione trasformarsi da vittima in carnefice? No, noi non siamo sicuri di questo. Sicuramente è positivo quanto è contenuto e quanto è previsto nel testo del disegno di legge; sicuramente è positivo il non dovuto risarcimento all'aggressore, che ha rappresentato il danno e la beffa più clamorosa che la giurisprudenza possa immaginare. Però voglio dire e voglio sottolineare con convinzione, da parte di Fratelli d'Italia, che concettualmente e direi ontologicamente questo provvedimento doveva e voleva fare di più. Lo dico perché sono convinta che, anche nell'animo di chi ha promosso per primo (dopo di noi) questa riforma, sicuramente non si è raggiunto quello che si è predicato e non si è raggiunto compiutamente quello che forse all'inizio ci sarebbe voluto. Noi infatti riteniamo che non sia concettualmente e ontologicamente declinato un principio fondamentale, che è il diritto e il dovere alla difesa quando si è vittima di un'aggressione. Se entri a casa mia, non mi interessa il motivo per cui entri; stai violando la mia casa, stai violando la mia famiglia e rappresenti una minaccia che non sono in grado di prevedere, la cui gravità non sono in grado di prevedere e che non devo

opposizione patriottica e responsabile e vorrei che la maggioranza prendesse atto che quando, come nel caso di ieri, presentiamo emendamenti per aiutare un provvedimento, forse ci vorrebbe più considerazione per chi si impegna comunque per il bene del Paese senza avere un pregiudizio nei confronti della maggioranza di Governo. Pertanto, rispetto al testo in esame, con le perplessità che ho cercato di illustrare a quest'Assemblea, voteremo comunque a favore, considerandolo un passo in avanti, ma non quanto si era promesso, perché per Fratelli d'Italia la difesa è sempre legittima, è un principio, è un diritto e questa legge, utile, buona, positiva, compilativa in alcuni aspetti, non rende la difesa sempre legittima.

Vorrei altresì dedicare un pensiero alle persone che hanno vissuto l'esperienza di doversi difendere prima da un'ingiusta aggressione e poi da un ingiusto processo *(Applausi dal Gruppo al benzinaio Graziano Stacchio, al gioielliere Robertino Zancan, a Franco Sicignano e alla memoria di Ermes Mattielli, morto di crepacuore a seguito del processo a suo carico.

proponeva di specificare che per essere legittimati alla difesa occorre che l'aggressore usi le armi e non solo minacci di usarle. di usarle. Se non ci fosse da piangere ci sarebbe da ridere, ma mi chiedo come si fa a dire cose simili. Seguendo questa logica, uno che si trovi un aggressore in casa potrebbe difendersi solo dopo aver ricevuto tre o quattro colpi di pistola, ma non mi risulta che i morti siano in grado di difendersi *(Applausi La verità è che il testo è equilibrato e le critiche provenienti da destra e da sinistra lo testimoniano. La legittima difesa sussiste sempre quando viene violata la sacralità della casa familiare, luogo in cui ciascuno di noi ha il diritto di sentirsi al sicuro.

Niente più condizionale agli aggressori che non pagano prima il risarcimento del danno; pene più gravi per chi aggredisce la sacralità della famiglia, ma soprattutto niente più processi civili assurdi contro le vittime che, dopo essersi dovute difendere, devono anche affrontare un processo civile di risarcimento del danno. L'altra significativa introduzione è quella del gratuito patrocinio, non già per gli imputati, ma finalmente per le vittime di queste aggressioni. Penso che questa norma fortemente voluta dalla maggioranza degli italiani sia una norma di semplice buonsenso. Concludo con le parole di un gigante del secolo scorso, San Giovanni Paolo II, il quale diceva che la legittima difesa può essere non soltanto un diritto, ma un grave dovere per chi è responsabile della vita altrui, del bene comune, della famiglia e della comunità civile. Oggi abbiamo realizzato questa profezia.

tanti emendamenti che avevamo presentato in Commissione e in Aula non sono stati approvati. Speravamo che il passaggio alla Camera ci rendesse giustizia, per adattare questo provvedimento alle alle esigenze che noi rappresentavamo con il disegno di legge che aveva come primo firmatario La Russa, sottoscritto da tutti i componenti del Gruppo al Senato: purtroppo questo non è avvenuto. Questa terza lettura si caratterizza soltanto per la norma finanziaria relativa al gratuito patrocinio. Noi voteremo a favore, perché sappiamo che è un passo in avanti; ma è un passo in avanti, come hanno chiaramente illustrato, anche sotto il profilo giuridico, sia il collega Balboni che la collega Rauti, che non ci soddisfa per l'obiettivo che volevamo raggiungere. Vi sono, infatti, due aspetti della della norma che fra poco approveremo che ci mettono nella difficoltà di dare corso a ciò che l'opinione pubblica ci chiede. Quando facciamo riferimento alla eccessiva discrezionalità del giudice, non lo facciamo perché riteniamo che non ci debba essere il controllo di legittimità sul comportamento di chi si difende a casa propria; noi lo sosteniamo perché riteniamo che sia diversa l'accezione concettuale del significato di difendersi a casa propria e quindi di non dover dimostrare il grave turbamento o la proporzionalità. È una presunzione

chi si difende perché aggredito a casa propria non può valutare, nel momento dell'offesa, se la sua difesa è proporzionata o no all'azione di chi si introduce furtivamente a casa sua. Vi è un secondo aspetto

non cambia minimamente la normativa sull'uso e sul controllo delle armi in Italia; come è stato detto dalla senatrice Rauti, non esiste in Italia una normativa pari a pari a quella che vi è in tante altre parti del mondo (si fa spesso riferimento agli Stati Uniti d'America) e non vi è alcun mutamento. L'Italia è una delle Nazioni con più restrizioni, anche dal punto di vista amministrativo,

al Senato abbiamo sentito tanti rappresentanti del mondo dell'imprenditoria e del commercio dire che il 93 per cento degli imprenditori non vuole usare le armi. Questa norma, quindi, serve soltanto a coloro i quali hanno la capacità e la volontà

nella possibilità di difendersi, anche questa norma possa entrare nel vivo della società italiana, in attesa di poterla modificare ulteriormente, a vantaggio di chi viene offeso a casa propria e vuole difendersi.

che credo di poter dire ci appartenga per una primazia in una battaglia, quella appunto sulla legittima difesa, che va nell'ordine di salvaguardare la sicurezza del popolo italiano. La *ratio* di questa norma non è infatti quella di fare più morti e non è quella di togliere la vita a qualcuno, perché quando si viene aggrediti nella propria abitazione non esiste l'*animus necandi* e non c'è la volontà

di questa norma e non solamente di alcune categorie che certamente sono le più bersagliate, ma la sicurezza di tutti: la sicurezza anche di coloro che non si possono permettere di avere un allarme in casa o di avere la polizia privata che li controlla; la sicurezza di chi, Presidente, vive in condizioni di disagio e magari deve difendere un minimo di patrimonio che ha raccolto con enormi difficoltà, attraverso il lavoro, la fatica e il sudore della propria fronte. Ecco perché

alla violenza si può rispondere legittimamente con una violenza in senso positivo. Questo è il motivo per il quale voteremo a favore di questo provvedimento, in considerazione anche di un altro

abbiamo la consapevolezza che una buona parte di costoro delinquono. Non lo diciamo semplicemente noi, ma lo dice la cronaca dei giornali, lo dicono le statistiche giudiziarie e lo dicono i procuratori della Repubblica. Vorrei ricordare quello che ha dichiarato il procuratore generale della Repubblica di Bologna presso la corte d'appello, Ignazio De Francisci, nell'ultima relazione del 2018: «L'Italia non è solo diventata un Paese importatore di detenuti stranieri, che preferiscono il nostro sistema a quello del loro Paese, ma diventerà ben presto una sorta di paradiso penale per i latitanti rumeni e di tutti gli altri Paesi dell'Est». Accade spesso che l'arrestato rumeno, quando si dà esecuzione a un mandato di arresto europeo, venga rimesso in libertà, in quanto la Romania o non risponde alle richieste di informazioni sullo stato delle sue carceri, o prende addirittura tempo. Abbiamo in Italia bande di delinquenti efferati che provengono dall'Est che consumano violenze inenarrabili, spesso nei confronti di anziani, di persone giovani e di coloro che si trovano in uno stato di minorata difesa. Noi abbiamo l'obbligo e il dovere giuridico di intervenire pesantemente con una norma che possa davvero dare

ci hanno abituato ormai da troppo tempo certe sentenze, che potremmo definire arcobaleno o addirittura con altri termini, che hanno messo in difficoltà lo stesso ordinamento. Si tratta di sentenze creative, nelle quali

attengono alla cultura del popolo italiano, e noi difendiamo, in questa situazione, la vita e la proprietà: questo è il nostro obiettivo.

evitare, in tantissimi casi, quella graticola giudiziaria che trascina l'imputato che si è difeso per troppi anni davanti ai tribunali. Questa deve essere la nostra impostazione. Ecco perché la norma in fondo non fa

coloro che ci hanno aggredito - o eventualmente la procura della Repubblica - a dover dimostrare che c'è una sorta di responsabilità. Quando vengono i clienti, anche nel mio studio, in alcune occasioni sono persone che si ritrovano a dover rispondere di eccesso colposo in legittima difesa o anche di omicidio. Mi domando

difesi. In tantissimi casi si dice che è meglio la voce severa del magistrato rispetto a quella soave e consolatoria del sacerdote. In tantissimi casi ci si difende da situazioni realmente drammatiche. Noi abbiamo la convinzione che in uno Stato di diritto si debbano preservare anzitutto coloro che vengono aggrediti.

Sono situazioni particolarmente delicate e drammatiche, però ricordiamoci anche che in Italia il numero di coloro che detengono le armi è estremamente esiguo:

entrare all'interno delle nostre case, calandosi come la befana giù per il camino, oppure arrampicandosi come acrobati sui muri, sfondando le porte e usando la violenza, dobbiamo ricordare a costoro che può esserci anche un'altra alternativa. Ci sono mestieri che hanno dei rischi; se faccio l'imprenditore posso fallire; se faccio il chirurgo e dimentico il bisturi nella pancia di qualcuno, sicuramente rischio un'azione di risarcimento e l'apertura di un procedimento penale.

con i presupposti per l'esercizio della scriminante, cioè della non punibilità del fatto, e, poi, il secondo, terzo e quarto comma che modificano la portata della difesa nell'ambito del domicilio o di luoghi che siano assimilabili ad esso o alla privata dimora.

Gli aspetti positivi sono stati già messi in evidenza. Innanzitutto chi si difende dopo anni di processo e vede riconosciuta la

e cioè che la cosiddetta concezione liberale presuppone che lo Stato sia la derivazione del *pactum subiectionis* dei cittadini, che danno allo Stato il riconoscimento del proprio diritto e ricevono in cambio tutela. Per avere questo, sacrificano parzialmente il diritto di libertà, di proprietà e i diritti individuali. per questa ragione noi abbiamo insistito e richiesto che il provvedimento sancisse il diritto di difesa, che recava con sé una conseguenza evidente: chi agisce nel diritto di difesa, non è punibile per un fatto

in luce anche negli interventi di questa mattina, perché evidentemente, nella cornice che opera nell'ambito dell'articolo 52, le modifiche che abbiamo apportato all'articolo 2044 del codice civile sono parziali. Rimane infatti il dovere della cosiddetta indennità,

Il relatore Ostellari lo sa bene, perché in Commissione Forza Italia è stata chiarissima sul punto, ponendo la questione con specifici emendamenti. C'è una discrasia in ciò, in quanto la non punibilità penale rimane e residua dal punto di vista delle conseguenze civilistiche degli effetti. L'hanno già detto i miei colleghi: Forza Italia voterà a favore di questo provvedimento, anche se non è quello che avremmo voluto, perché avrebbe dovuto spiegare un concetto diverso: la difesa non è una scriminante, ma un diritto.

credevo veramente che oggi non ci fossero differenze e distinzioni su questo provvedimento, convinta che una parte della politica - soprattutto la sinistra avesse abbandonato il proprio atteggiamento ideologico quando si parla di sicurezza e riuscisse a capire ciò di cui i cittadini italiani hanno bisogno noi sappiamo benissimo. Basta andare in giro per le strade delle nostre periferie e in tutti i quartieri, infatti, per capire che essi vogliono che difendersi sia un diritto e che la difesa sia sempre legittima.

da Fratelli d'Italia alla Lega, a Forza Italia - avevano detto in campagna elettorale. Fermo restando che questa legge è un passo in avanti rispetto alla precedente e che Fratelli d'Italia è assolutamente d'accordo, ci aspettavamo però più coraggio dagli amici della Lega, perché ci sono cose che avrebbero potuto essere diverse, come la questione del turbamento emotivo, che ancora esiste.

Peccato per chi, vedendo queste discussioni, percepisca il disinteresse di moltissimi colleghi, perché qui stiamo parlando di un tema dirimente per la sicurezza degli italiani,

perché rimane la questione del turbamento emotivo. Ritengo molto difficile avere il termometro del turbamento emotivo di un individuo dopo che ha commesso un'azione,

entrasse nelle nostre case, non certo per venire a prendere il tè con i pasticcini, credo che la nostra adrenalina e il nostro turbamento emotivo sarebbero a livelli altissimi, perché lo spavento e la paura che possa succedere qualcosa ai nostri cari

Ritengo che il principio della legittima difesa debba essere un diritto, perché tutti dovremmo poter difendere i nostri cari e le nostre cose in qualsiasi momento,

per capirlo - che la paura sta aumentando; anzi stiamo correndo un pericolo perché stiamo passando dalla paura all'ostilità. Gli italiani diventano ostili, perché non si sentono sicuri nelle proprie abitazioni.

abbia sicuramente il favore della maggioranza dei cittadini italiani. È una legge che cambia, nella sostanza e in profondità, quello che era prima e che consentirà

per far del male e rubare. Tutto questo non ci sarà più ed è per tale ragione che noi siamo favorevoli al

a riprendere in mano un provvedimento che avrebbe meritato, anche in sede di prima lettura alla Camera, ben altra attenzione e non semplicemente un aggiustamento della vicenda economica relativa all'anno passato. Avrebbe meritato più attenzione, avrebbe meritato aggiustamenti, avrebbe dovuto riportarci nell'alveo della legalità e della legittimità, perché oggettivamente non si può condividere quello che è stato detto negli interventi che mi hanno preceduto, perché si sta stravolgendo un sistema. si sta stravolgendo un sistema. Oggi finalmente si è avuto il coraggio di parlare - lo stesso relatore l'ha fatto - della minaccia che nascerebbe dall'introduzione di taluno nell'altrui abitazione contro la volontà del proprietario ed è quello che ci siamo attardati a dire mille volte durante la discussione - che peraltro spesso era un soliloquio - in Commissione, una discussione che non prodotto praticamente niente, perché ormai si sta andando avanti con un attacco al parlamentarismo che ormai è evidente e sotto gli occhi di tutti. È un attacco che non consente di fatto di confrontarsi in maniera corretta, non consente, nell'ambito dei lavori di Commissione e di Assemblea di avere un confronto serrato, di cercare di capire quali sono

il contenuto delle audizioni che ci sono state. Stamattina però ho sentito dire da qualcuno che questo provvedimento ha accolto le indicazioni che erano pervenute dai soggetti auditi. Ebbene, io sono mediamente distratto, ma francamente non arrivo ad essere distratto fino a questo punto, perché i soggetti auditi hanno detto esattamente il contrario. soggetti auditi si è detto d'accordo con il contenuto di questo provvedimento, mentre tutti gli altri (magistrati e avvocati) si sono detti contrari al mutamento di un sistema che era oggettivamente corretto e che forse avrebbe avuto bisogno di qualche aggiustamento nel concetto dell'eccesso di legittima difesa. Tutti i soggetti auditi hanno detto questo e infatti noi stessi avevamo proposto una modifica al concetto dell'eccesso colposo di legittima difesa e pensavamo che con quello si potesse chiudere. Così non è stato,

era il caso di consentire l'utilizzo delle armi. Hanno fatto presente che quei soggetti sensibili che si trovano ad essere aggrediti, pur essendo armati, hanno delle difficoltà oggettive a sparare contro un essere umano; hanno detto che non erano capaci di fronteggiare l'assalto di quelli che invece arrivano consapevoli del rischio che corrono e quindi pronti anche all'uso delle armi. Nessuno però ha chiesto di essere

prevedeva e fino ad oggi prevede il criterio di proporzionalità tra offesa e difesa. Questo criterio di proporzionalità oggi viene di fatto buttato alle ortiche e si introduce la possibilità di sempre contro chiunque si introduca, anche per errore (lo abbiamo detto mille volte nel corso della discussione), nell'abitazione altrui. Sono stati fatti degli esempi, li ho fatti io e li ha fatti molto meglio di me il senatore Grasso, che ha detto che in questo modo stiamo autorizzando a sparare anche nei confronti del vicino di casa che si introduce nel giardino per raccogliere la palla che ha perso il bambino o nei confronti del figlio che esce, magari di nascosto, di notte e si dimentica le chiavi a casa ed entra dalla finestra: si consente di uccidere in queste condizioni per un mero errore. Inizialmente, addirittura, si era arrivati alla aberrazione che non fosse possibile neanche la valutazione da parte del giudice: è legittima difesa e rimane legittima difesa. Poi fortunatamente ci si è resi conto - anche per le indicazioni che sono pervenute da soggetti auditi, che hanno detto che il controllo del giudice è necessario per stabilire se effettivamente sussista o no la legittima difesa, perché altrimenti si correrebbe il rischio di coprire addirittura gli omicidi volontari - che a questo non si poteva arrivare. arrivare. Si sta tentando, semplicemente, di fare l'ennesimo *spot* elettorale con la forza dei numeri. A questi numeri ci dobbiamo piegare, ovviamente, ma la nostra voce abbiamo il dovere di farla sentire, a difesa dei princìpi democratici che fino ad oggi hanno ispirato l'attività giudiziaria di questo Paese: quei princìpi di giustizia che sono connaturati nel nostro sistema. Purtroppo, però, tutti gli emendamenti che abbiamo proposto sono stati ritualmente respinti. Voglio, però, sottolineare anche un altro aspetto,

era stata sempre concertata con i soggetti protagonisti, cioè con il personale amministrativo, con i magistrati e con gli avvocati, con i quali si è vantato di avere un confronto assiduo e continuo.

l'esito delle audizioni e ve ne renderete conto. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Nel corso di quelle audizioni è stato detto in maniera chiarissima che il sistema va bene così com'è. Lo ribadisco, l'unica cosa cui si poteva mettere mano era l'eccesso colposo in legittima difesa. Invece no. Oggi, con uno *spot*, che è semplicemente e ancora una volta una *captatio benevolentiae* e una ricerca di voti, si è detto: «No, d'ora in avanti, se qualcuno vi offende, tranquilli, vi potete difendere, potete sparare». È stato detto anche stamattina in quest'Aula. Siamo all'aberrazione giuridica. Ora, non è questo il primo provvedimento nel quale l'esito delle audizioni viene regolarmente disatteso; talvolta ci viene anche da pensare che siano totalmente inutili, perché ormai si è preso questo abbrivo: non si discute più nulla, arrivano i provvedimenti del Governo, vengono "scodellati" e non si possono modificare. Questo accade regolarmente. La discussione è il più delle volte mortificata e, consentitemi di dirlo, questo è palesemente un attacco al sistema parlamentare che - vivaddio - fino ad oggi è stato uno dei cardini del nostro sistema democratico. Si vuole apparire come salvatori della Patria e talvolta si indossa la divisa per dire che si vuole essere garanti della giustizia giusta, ma, in effetti, tutto questo è soltanto apparenza. C'è la volontà di imporre le proprie idee, che troppo spesso violano palesemente i princìpi basilari del sistema democratico, i princìpi basilari della democrazia, i princìpi basilari dell'uguaglianza, i princìpi basilari del diritto alla vita, in questo caso specifico,

anche ieri, a riprova di quanto ho appena detto (vale a dire che il nostro sistema con gli *spot* elettorali sta andando a farsi benedire), è nuovamente emerso che le carceri sono sovraffollate. Si badi bene: sono sovraffollate non perché siano aumentati gli arresti, che invece sono diminuiti, ma perché si sta attaccando, come dicevo, quel sistema fondato sulle libertà dell'individuo, fondato sul riconoscimento della dignità dell'uomo, dignità che è anche di coloro che vengono incarcerati per aver sbagliato i percorsi di vita.

infatti, è fondato sull'imposizione da parte di un Governo che tende a limitare i diritti dell'individuo e, in questo caso, sta armando persone che,

favorire l'autodifesa, che porterà sicuramente, come dicevo, ai risultati di cui ho parlato. Quando inizieranno a vedersi i morti,

sparare contro queste persone, allora cominceremo a dire che forse abbiamo sbagliato qualcosa e forse sarà opportuno tornare indietro. Noi - ricordatelo - ve l'avevamo detto.

da tanti anni, da tanto tempo, il Paese e i cittadini chiedevano una risposta in termini di giustizia e in termini di sicurezza: in termini di giustizia per evitare processi ingiusti

domanda è rimasta inascoltata. La politica ha fatto finta di niente - e le istituzioni anche - e laddove invece ha prestato ascolto ha fatto qualche danno perché magari, per poter proteggere i propri cari e il proprio posto di lavoro, un cittadino aveva bisogno del metro per verificare se il ladro fosse un centimetro più in là o più in qua dell'uscio, oppure dell'orologio per vedere quanti minuti mancavano al tramonto e nel frattempo il danno sarebbe stato fatto. una risposta che, come diceva il nostro relatore, è equilibrata, una risposta che viene fuori dalle istanze parlamentari e che collima con l'esigenza di buon senso che emerge dal Paese. Vorrei parlare rapidamente di tre verità, o di tre bugie a seconda dei punti di vista. Innanzitutto, la legge che verrà approvata

luogo, non è vero che questa legge garantirà a prescindere l'impunità di chi sarà costretto a difendere la sua proprietà, la propria persona o i propri cari essendo obbligatoria, sarà avviata. Saranno avviate le indagini ma probabilmente, se il soggetto ha agito in uno stato di legittima difesa, tali indagini saranno prontamente archiviate e quindi non ci sarà un calvario per chi ha subìto già un danno perché questa legge pone delle regole certe e chiare. In terzo luogo, questa legge non sostituirà i cittadini allo Stato. È una legge che invece crea una simbiosi giusta tra istituzioni e cittadini. Lo Stato, purtroppo, non può essere ovunque, non può essere dappertutto in maniera celere e vi è la necessità, in tante circostanze, che un cittadino, nell'immediatezza di un fatto, possa poter difendere ciò che di più caro ha al mondo.

come cittadino, come imprenditore o come lavoratore nella propria casa o sul proprio posto di lavoro non può aspettare che un intervento dello Stato, seppur celere ed efficace,

Devo dire però che, nel frattempo, c'era stata una lunga discussione all'interno di Forza Italia, che ci aveva portato ad andare al di là della nostra primigenia proposta di legge. Per quanto mi riguarda,

ma questo non toglierà al giudice la possibilità e la facoltà di interpretare la norma e di valutare la situazione concreta che gli si presenterà, al fine di inquadrare penalmente la fattispecie

nei casi in cui sono superati i limiti dell'eccesso colposo, è giustificato e non può essere punito colui che abbia reagito in quelle condizioni.

ha suggerito di usare il termine «turbamento», prendendo spunto da quell'indicazione del nostro testo, ed essenzialmente di formulare l'articolo 55, comma 2, come un'ipotesi di lecito eccesso colposo.

rappresenta un dato formidabile: se è lecito, non ci può essere una responsabilità penale, ma non ci può essere nemmeno una responsabilità civile, perché a un comportamento lecito non può conseguire un addebito di responsabilità.

introducendo un indennizzo. Caro Pillon, ci sarà il processo civile, perché è il giudice civile che dovrà stabilire l'indennizzo. A

Eh no! Il danneggiato qui è l'aggressore, è colui che è entrato in casa nottetempo e che è stato ferito o ammazzato per una reazione di colui che stava in quella casa; in quel caso spetta l'indennizzo. Si apre quindi un lungo processo civile, che sostituisce il tempo del processo penale.

per avere la certezza di quanto dovrà pagare il povero Cristo che ha subito l'aggressione in casa. Il nostro voto a favore è dovuto al fatto che si tratta di un passo in avanti

una nuova filosofia di interpretazione del diritto penale ed è necessario sanzionare comportamenti che sono in contrasto con i princìpi costituzionali. Mi auguro che ci sia questa volontà, perché stiamo facendo molte leggi, con l'intenzione che dobbiamo sempre rimodularle e riconfermarle. Mi meraviglia e mi dispiace che non ci sia il ministro Salvini, perché aveva garantito la sua presenza in questa seduta (ma so benissimo che lui è molto attento e comunque gli si può riferire alla sua capacità, non dico di cambiare idea, ma di modulare l'intervento dello Stato in relazione alle necessità e alle interpretazioni che sorgono dalle leggi;

sulla percezione della sicurezza. Badate che questa norma non incide sulla sicurezza; il bisogno di sicurezza che c'è nel nostro Paese va risolto con alcune norme che il Ministro dell'interno dovrà portare, al fine di garantire quella sicurezza cui i cittadini hanno diritto. Questa norma incide sulla percezione della sicurezza,

con la lamentela di quanti avranno dovuto subire un lungo processo civile, che diranno di essere esposti a ulteriori conseguenze.

legge che ci apprestiamo ad approvare oggi è uno di quelli che hanno una ricaduta diretta sulla percezione dei nostri cittadini. Purtroppo tutti noi in quest'Aula possiamo dire di aver avuto notizia di un fatto grave accaduto vicino a noi,

A noi italiani è stata sottratta gran parte di quella cultura dell'accoglienza, facendo credere che sia appannaggio soltanto di una forza politica. Desidero spiegarmi meglio, perché secondo me questo è un concetto molto importante.

causa delle citate politiche scellerate del Partito Democratico, ad affrontare questi fatti in maniera drammatica ed emergenziale. Vorrei dire chiaramente che anche in questa maggioranza, checché se ne possa dire, è possibile trovare un atteggiamento di naturale tolleranza e attenzione verso determinate problematiche. *(Applausi In questo senso la politica disastrosa del Partito Democratico nell'accoglienza e nell'integrazione sociale ha completamente distorto la percezione delle comunità di cittadini italiani, che sono state portate all'esasperazione dalla incapacità della classe dirigente del Partito Democratico; pertanto ritengo giusto per questa maggioranza e ovviamente per gli italiani rivendicare una naturale, sostenibile e sana politica dell'accoglienza, fatta su numeri e soggetti che rientrino in un perimetro di legalità e sostenibilità.

si sono consumati almeno tre dei crimini più efferati della storia repubblicana dell'Umbria. E purtroppo, non da ultimo, nelle scorse settimane, nella mia città di origine, Spoleto, si è verificato un altro episodio grave di violenza domestica, perpetrata da criminali a seguito di una effrazione. Questi sono soltanto degli esempi, ma ciascuno di noi potrebbe fare lo stesso discorso. Sto parlando, signori, di omicidi commessi sull'uscio di casa: una coppia di anziani massacrata sul proprio letto; un giovane trentenne ternano letteralmente sgozzato all'uscita di un locale pubblico. Non è soltanto di fronte a questi fatti, ma è anche pensando ai nostri genitori anziani da soli a casa, o o magari a noi stessi e ai nostri figli o ai nostri amici, parenti o vicini, che possiamo dire che finalmente è arrivato il momento di considerare la difesa all'interno delle mura della propria casa o delle attività commerciali o imprenditoriali sempre legittima,

privata senza che ciò possa minimamente scalfire la salute, la psiche e lo stato d'animo di una persona. Voglio ripetere questo concetto contrario a quello che pensano gli intellettuali che hanno distrutto il nostro Paese, che ritengono legittimo introdursi all'interno di una proprietà privata, senza che ciò possa minimamente scalfire la salute, la psiche e lo stato d'animo di una persona. È chiaro che per quelli che noi abbiamo definito i "politicanti delle ZTL", che non frequentano le periferie, è difficile comprendere davvero cosa significhi integrazione nel degrado: è molto facile fare integrazione nei vostri quartieri agiati, è molto difficile farla nelle periferie periferie delle nostre città. Da oggi finalmente sarà possibile difendersi senza la preoccupazione di doversi a propria volta difendere da accuse di illegittima difesa. Finalmente viene meno anche la punibilità in sede civile, perché un'assoluzione in sede penale non corrisponderà necessariamente al risarcimento del danno derivante dal fatto. Pertanto, concludo il mio intervento ribadendo con forza il mio sostegno a questa iniziativa del Governo del cambiamento.

L'eccesso colposo oggi è punito penalmente e determina un risarcimento del danno; da domani l'eccesso colposo non sarà più punito dallo Stato e non darà più alcuna facoltà al soggetto che aggredisce di avanzare richieste di risarcimento del danno. Questo è chiaro nel testo. Gli interventi effettuati sono stati mirati non solo, ovviamente, alla legittima difesa, ma anche all'eccesso colposo ed a tanti altri argomenti (gli articoli sono nove

il senatore Cucca, la proporzione si presume sempre esistente, ovviamente se ci si difende da un'aggressione di quel tipo. Non abbiamo legittimato,

Senatore Cucca, ricordo che già nel 2006 qualcuno lo aveva detto,

Sono le stesse cose che si dicono oggi, in un clima che a mio avviso forse avete causato voi

Signor Presidente, ho ascoltato tutti e cercherò di rispondere in via generale. A cosa punta questa riforma? Punta all'ampliamento dell'applicazione della legittima difesa, all'inasprimento delle sanzioni per i reati di furto, violazione di domicilio e rapina e all'introduzione di una presunzione di legittima difesa domestica. Ci sono punti qualificanti nel disegno di legge. In estrema sintesi, possiamo dire che agisce sempre in stato di legittima difesa chi si trovi a dover rispondere a una intrusione violenta, nel proprio domicilio o nei luoghi di lavoro, compiuta con armi o con altri mezzi offensivi. Chi è aggredito, infatti, deve essere consapevole di poter reagire all'attacco senza dover temere un estenuante calvario giudiziario a proprio carico. Non sussiste, dunque, alcuna possibilità che la nuova norma possa essere scambiata per una licenza di uccidere, come qualcuno ha volutamente travisato. Al contrario, si elimina *ex ante* qualunque dubbio sul perimetro della condotta giudicata non punibile. Viene quindi allargata la tutela per la persona che reagisce per difendersi, mentre si riduce la discrezionalità a disposizione dell'autorità giudiziaria per valutare la legittimità dell'atto di difesa. Rimane l'eccesso colposo, ma viene introdotto anche il concetto di «grave turbamento» determinato dal pericolo in atto. In coerenza con queste previsioni della norma, chi si è difeso secondo quanto previsto dalla legge non dovrà pagare alcun risarcimento nel caso abbia provocato danni a chi l'ha aggredito. Infine, il patrocinio gratuito: chi si è difeso legittimamente da un attacco violento potrà beneficiare, durante il successivo procedimento penale, del patrocinio legale a spese dello Stato. Si tratta dunque di una di una riforma di buon senso, un passo in avanti nella civiltà del diritto perché punta a impedire il ripetersi di gravi ingiustizie. Non è infatti concepibile che chi si difende legittimamente da un attacco violento diventi vittima due volte, del criminale e poi dello Stato. Non una riforma di parte, ma di buon senso e secondo giustizia. Una norma a favore di tutti. Chi è aggredito deve potersi difendere, consapevole del fatto che non sarà vittima, oltre che dell'aggressione, anche di percorsi giudiziari lunghi e costosi, talvolta vere e proprie persecuzioni dall'esito incerto perché collegate a una troppo accentuata discrezionalità. Chi aggredisce e chi si difende non sono sullo stesso piano: da una parte c'è chi delinque, consapevole di correre dei rischi, dall'altra persone oneste che si oppongono al criminale che irrompe nelle loro abitazioni per rapinare, aggredire, picchiare o, peggio ancora, violentare. Noi siamo dalla parte dell'aggredito che legittimamente si difende. Non c'è dubbio che la maggioranza degli italiani sia convinta che, in questi anni, sia prevalso un pregiudizio nel giudicare molti di questi casi, tutti a sfavore dell'aggredito e a tutela dell'aggressore.

per i preziosi contributi e per l'impegno preso con gli italiani e oggi rispettato.

la provocazione - se volete, l'annotazione - che ho appena ascoltato da parte del senatore Lucidi, che è intervenuto in discussione generale, perché ha detto una cosa che in fondo condivido. Secondo in questo strano Paese, nella discussione pubblica, nel dibattito politico, accade che si inneschi un meccanismo per cui sembra ci siano temi - di fatto spesso è così - appannaggio della sinistra. Lucidi faceva riferimento al tema dell'immigrazione, salvo poi, in alcuni passaggi, aver trattato quel tema in un modo diverso da come ci si aspettava.

quell'altro campo politico, appunto, quello che sento personalmente molto distante, persino opposto da me, e cioè la destra. È la destra che si occupa di sicurezza, e devo dire che tra le cose da sanare c'è anche un ritardo, per quanto ci riguarda, nell'affrontare un tema delicato che ha a che fare spesso con i soggetti più deboli. È ai soggetti più fragili che bisogna garantire un di più di sicurezza, e su questo c'è un lungo lavoro da fare. Il tema, signor Presidente, se la destra si stia occupando esattamente di questo o, per l'ennesima volta, stia mettendo in campo una grande operazione propagandistica. Lo dico ai colleghi ai colleghi presenti in questa Aula per il suo tramite; vorrei dare una notizia che non lo è: la legittima difesa esiste

chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa». del pericolo di un'offesa e l'ordinamento prevede già la possibilità di difendersi in una situazione in cui il soggetto si sente minacciato o ha la percezione di sentirsi minacciato da questo pericolo. Peraltro,

della propria o altrui incolumità, aggiungendo la difesa dei beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. Siamo di fronte al fatto che,

della legislazione introdurrà elementi di incertezza che mineranno la sicurezza dei cittadini e non il contrario. Questa è la prima notazione. La seconda: vi pare che su un tema così delicato così delicato si sia voluta inserire una veste normativa a concetti di natura soggettiva, come il turbamento? Siamo nella sfera

chi è più soggetto a *shock* di carattere emotivo oppure addirittura chi è più disponibile per animo a reazioni incontrollate, è più nelle condizioni di dover reagire con un'arma di difesa? E deve essere giustificato per questa ragione? Stiamo parlando di questo? State introducendo un elemento di incertezza non

che modifica l'articolo 165 del codice penale in materia di obblighi del condannato. Se passa infatti la formulazione, nel caso di condanna per furto in abitazione o con strappo, per esempio, il beneficio della sospensione condizionale della pena sarebbe sempre e comunque subordinato ad un requisito economico. Sostanzialmente solo chi si può permettere il risarcimento può accedere al beneficio della sospensione

strettamente legislativo o giuridico, ma tutto politico: inserire un meccanismo automatico e deterministico e sottrarre alla discrezionalità del giudice, l'unico che ha in mano gli elementi per fare una valutazione, anche riguardante la sfera più

rappresenta - abdichi sostanzialmente alla propria funzione, ossia garantire la sicurezza dei propri cittadini. Egli dice dunque ai propri cittadini: siccome non sono in grado di mettere in campo politiche di prevenzione

non solo il lume della ragione, ma l'occasione di rafforzare lo Stato di diritto, perché in realtà questa roba qui, la schifezza che state facendo, lo facendo, lo rendono più fragile. È qualcosa di assolutamente insostenibile e insopportabile, rispetto alla quale esprimiamo tutta la nostra contrarietà, che naturalmente non si fermerà con questo voto, ma che porteremo anche fuori dal Palazzo.

coloro che ci hanno mandato qui e che abbiamo il dovere di ascoltare. Già nel 2006 la normativa della legittima difesa, che era andata bene per tanti anni,

venivano commessi furti in casa, per cui i ladri stavano attenti a verificare quando non vi fosse nessuno e poi compivano la loro opera delinquenziale. L'immigrazione dall'Est ha portato in Italia una metodologia

se ne va con il bottino e, spesso, con la vita del derubato. Questa nuova realtà, di fronte alla quale la sinistra ha gli occhi bendati, ha portato alla necessità di offrire alla magistratura una legge che ne tenesse conto. È colpa nostra se nel 2006 non abbiamo saputo fornire una normativa chiara

lasciava libero spazio alla discrezionalità e alla diversità di giudizio da magistrato a magistrato. Pertanto, come testimonia il fascicolo che avete in mano, noi

di detenzione di armi; anzi, la vostra predicazione del *far west,* falsa e bugiarda, ha portato a una cosa incredibile:

desistenza e pericolo di aggressione. È giusto che per difendersi si debba controllare che vi sia un pericolo di aggressione, ma davvero, cari colleghi, avete fatto bene a respingere il nostro emendamento che voleva eliminare l'analisi della desistenza da parte dell'aggredito? Davvero pensate che chi a casa propria trova una persona che sta entrando in maniera violenta

È sbagliato aver respinto questo emendamento, così come sbagliato è stato insistere sul fatto che il turbamento debba essere grave, è un'altra discrezionalità che mette in imbarazzo la magistratura. Sarebbe bastato parlare di turbamento. Quand'è che un turbamento è grave e quand'è che non è grave? Chi lo decide?

di questa norma, che avremmo voluto correggere con i nostri tre emendamenti, compreso quello sull'arma legittimamente detenuta, che non avete voluto correggere. Ci va bene lo stesso. È comunque un passo avanti nella difesa e nella tutela

di trovarsi sotto il fuoco di un delinquente nella propria abitazione o sotto la minaccia della propria incolumità di notte o di giorno, ha poi subìto propria pelle l'onta di un processo e qualche volta di una condanna, ma basta anche un'assoluzione che arriva dopo tre anni per essere un male - questo sì - ingiusto, che noi abbiamo sempre cercato di eliminare. Parlando solo dei lombardi, dedichiamo questo nostro voto a Mario Cattaneo di Casaletto Lodigiano, a Rodolfo Corazzo di Rodano, a Francesco Sicignano di Vaprio D'Adda e a tutti gli altri aggrediti ingiustamente perseguitati da uno Stato fino adesso cieco, che grazie a questa legge mi auguro non lo sarà più. Signor Presidente, in un recente dibattito televisivo ho sentito alcuni esponenti del MoVimento 5 Stelle sostenere che la questione della cittadinanza ai bambini che nascono in Italia da coppie straniere non è una priorità. Io trovo che sia un'opinione legittima, ma che sia un'opinione espressa in un Paese in cui 70.000 bambini l'anno nascono da coppie straniere. Mi domando però perché, allora, in questi anni è diventata una priorità la legittima difesa, questione assolutamente marginale. Negli ultimi dieci anni non sono mai stati più di dieci l'anno i procedimenti per abuso o abuso colposo di legittima difesa. allora diventa un tema su cui mobilitare l'informazione, le Camere, il lavoro del Parlamento? La risposta è semplice: si usa la questione per cavalcare paure legittime e fare propaganda per mascherare l'incapacità di rispondere alla domanda di sicurezza che c'è nel Paese. Questa è una legge che cancella uno dei fondamenti della nostra Costituzione e dello Stato di diritto, quello della proporzionalità tra offesa e reazione difensiva. La legge dice infatti che la reazione difensiva è sempre *a priori* proporzionata e quindi si può sparare a una persona che sta scappando dopo essere stata scoperta o solo perché si trova all'interno del proprio giardino. Nonostante ci abbiate provato, non siete riusciti però ad evitare che comunque ci sia una valutazione da parte della magistratura, ma cancellare il principio di proporzionalità è un'aberrazione. Come abbiamo già dimostrato nella scorsa legislatura, noi condividiamo la necessità di stare a fianco delle vittime di reato che sono state costrette a difendersi, arrivando a introdurre il concetto di grave turbamento e riconoscendo il risarcimento delle spese processuali per chi si è difeso legittimamente, ma cancellare il principio di proporzionalità cambia tutto. Mi Mi preoccupa questo principio di proporzionalità cancellato, se associato a un'affermazione che il Ministro dell'interno ripete spesso quando siamo di fronte a episodi di questo tipo: se la sono cercata. Quel «se la sono cercata» giustifica qualunque comportamento? Quel «se la sono cercata» che cosa vuol dire? Che si può fare qualunque cosa a una persona che se lo sia meritato? Non c'è alcuna pietà umana, non c'è alcuna valutazione sul valore di una vita umana. «Se la sono cercata» non può essere una categoria che usano le istituzioni. Non può esserlo. La pericolosità di questo provvedimento sta qui. Non sta solo nel merito, ma nel messaggio che incentiva i cittadini a difendersi da soli e che propone un modello di società pericoloso. Questo provvedimento, associato a quello che avete voluto e che ha recepito in modo estensivo la direttiva europea sulle armi, consentendo la libera vendita di armi più pericolose di quelle che erano consentite prima e riducendo i requisiti per l'acquisto, rischia di aprire una strada a quella cultura che mi pare sia il riferimento di molti degli argomenti che ho sentito cultura che ha portato i Paesi che hanno adottato questa linea, come gli Stati Uniti, a contare nel 2017 40.000 morti uccisi da armi da fuoco. In un anno solo, due terzi dei morti che ci sono stati nel Vietnam. Tenete conto che l'Italia, già oggi, è il primo Paese per morti ammazzati da armi da fuoco in Europa, nonostante siamo il quindicesimo per armi possedute. dal Gruppo PD)*. Ho detto che questa legge interviene su una questione marginale. Negli ultimi anni i processi per abuso di legittima difesa o abuso colposo sono stati pochissimi. E ciò rende evidente che ciò che conta per voi, per chi l'ha proposta, sono i messaggi potenti e dannosi che volete trasmettere: armatevi per difendervi, perché le istituzioni non sono in grado di tutelare le persone. Questo è il messaggio. Non solo non c'è più sicurezza dopo questo manifesto sulla legittima difesa, anzi, i cittadini si sentiranno più soli e abbandonati a se stessi da un Governo che, anziché investire per rendere più sicure le nostre città, preferisce alimentare le paure e dire: difendetevi da soli Noi non siamo capaci di garantire la sicurezza. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Il fatto che sia il Ministro dell'interno e non quello della giustizia a intestarsi questa norma la dice lunga. Chi deve garantire sicurezza dà ai cittadini un messaggio di impotenza. Dice: fate voi, arrangiatevi. Noi ve lo consentiamo. E se questa scelta comporterà più vittime si dirà che se la sono cercata, come si dice troppo spesso, e chi se ne frega se stiamo parlando comunque di vite umane. È una bandiera ideologica. Oggi la approverete vedremo le conseguenze nei prossimi anni, ma due cose vanno dette. La prima: non ci sarà più sicurezza e i cittadini lo devono sapere. I casi qui citati, gli anziani uccisi mentre dormivano e altri casi, non si risolvono armando le persone o pensando che possano armarsi e difendersi da sole nelle case. come dimostra la storia dei Paesi che hanno adottato queste strategie, dove questa strada è stata intrapresa ci saranno più armi e ci saranno più morti. La seconda: vi assumete *in toto* la responsabilità di queste scelte. Non ve l'ha chiesto il popolo. Non è la legge che voleva il popolo. Ve lo state inventando. Il popolo non vuole la legge per potersi difendere da solo, come voi raccontate. Avete fatto di questa vicenda una bandiera ideologica. Le persone chiedono sicurezza e prevenzione, di non essere lasciate sole di fronte ai pericoli. A queste domande voi non sapete rispondere se non facendo credere loro che la soluzione è difendersi da soli. Voteremo no per queste ragioni. Voteremo no per questo manifesto ideologico. Voteremo no per una legge che diminuirà la sicurezza in questo Paese.

Nel provvedimento che votiamo oggi non c'è alcun riferimento alla licenza di uccidere, alcuna volontà di trasformare il Paese in un *far west*, di trasformare i nostri cittadini in pistoleri, né tanto meno di dare la possibilità di sparare alle spalle quando un ladro entra in casa tua.

dice solo fantasie che sono state create *ad hoc* per cercare di mettere in difficoltà, creare dei dissapori all'interno della maggioranza di Governo, tra le forze di Governo ma anche tra la maggioranza di Governo e la magistratura. Non è così. Questo è un provvedimento equilibrato, di buon senso, che sancisce un sacrosanto diritto che è quello di potersi sempre difendere in casa propria.

per violentare, per aggredire deve anche mettere in considerazione il fatto che può subirne le conseguenze, che corre un rischio. Dal provvedimento emerge chiaramente che vogliamo mettere in evidenza soprattutto il fatto che la tutela dell'aggredito deve prevalere sulla tutela dell'aggressore. La legge, infatti, prevede la non punibilità per chi agisce in stato di grave turbamento derivante da una situazione di pericolo e di chi agisce per difendere la propria e altrui incolumità. È una legge che serve per difendere le vittime, perché chi si è difeso, chi ha reagito, spesso e volentieri, poi, ha dovuto subire un vero e proprio calvario giudiziario. Tranquillizziamo tutti: non è vero che non ci saranno le indagini. Tutte le volte che ci sarà un'aggressione è evidente che le indagini ci saranno, quindi la magistratura il suo lavoro lo farà, come l'ha sempre fatto perché anche su questo punto sono state dette delle bugie e sono state espresse fantasie, sempre per alimentare tensioni che non era necessario alimentare. Le indagini ci saranno. Certo, qualcuno della minoranza sostiene che in realtà già oggi la legge sulla legittima difesa esiste e che in molti casi si è arrivati ad una in molti casi si è arrivati ad una assoluzione, ossia le persone che hanno reagito sono state poi dichiarate innocenti perché la magistratura ha verificato che non c'era eccesso colposo di legittima difesa.

questo non sarà più possibile perché le persone, se alla fine saranno dichiarate innocenti, non dovranno più pagare le spese legali, che saranno a carico dello Stato, com'è giusto che sia. modo, non ci sarà più la necessità di risarcire i malviventi, che è una delle cose più intollerabili

non siano stati accolti. Riteniamo che questa legge sia un passo in avanti, ma forse qualcuno ha dovuto frenare un po' per qualche alleato indeciso sui temi FI-BP)*. I tempi sono stati un po' lenti, non basta la scriminante. Noi vogliamo dire con chiarezza un sì al diritto alla difesa del cittadino e vogliamo dire anche no alla doppia aggressione. Vedete, sono stati citati in questi mesi tanti casi: ci sono persone che hanno subìto prima l'aggressione del criminale e poi l'aggressione di un giudizio durato fino a sei anni (un'ulteriore pena ingiusta). Ora questa legge non abolisce la valutazione del magistrato, ma sposta il baricentro dalla parte del cittadino aggredito. Si poteva fare, ministro Salvini, qualche passo in più in più e, lo faremo quando ci sarà omogeneità culturale e programmatica nelle forze di Governo. Ma questa - come si suol dire - è un'altra storia. La legge quindi è un deterrente, ma anche un avviso. Noi non vogliamo una Nazione armata. Che questa legge, però, ampliando i margini di azione e di difesa del cittadino, costituisca un deterrente nei confronti del crimine, non è un fatto negativo: la deterrenza delle norme è uno degli strumenti per garantire la legalità. E voglio ricordare non solo le persone come Stacchio e tante altre, che tutti abbiamo conosciuto in questi anni e che sono protagoniste vive di episodi di legittima difesa. Vorrei che quest'Aula ricordasse anche tutti quelli che invece sono morti tentando di difendersi, perché aggrediti dal crimine.

per il suo spirito, definimmo insufficienti; e purtroppo siamo ancora di questo avviso. Ci lamentiamo di ciò che si può fare in più e non si fa, e non di ciò che si fa su certi temi.

ovviamente con l'equilibrio necessario. Se fossero stati approvati i nostri emendamenti, avremmo avuto ancora più chiarezza; ci sono delle cadute civilistiche e nasceranno aspetti interpretativi, ma ci sarà tempo e modo di occuparsene. Voglio dire con chiarezza che questa non è una legge

Noi abbiamo detto fin dall'avvio di questa legislatura che avremmo difeso tutti gli argomenti tratti dal programma del centrodestra; peraltro, le proposte di Forza Italia anche qui in Senato sono stampate e documentate. Questo era uno dei princìpi cardine della politica della sicurezza che il centrodestra ha proposto e, quindi, noi siamo lì dove gli elettori

lavoro. Noi voteremo a favore, consci della battaglia che abbiamo condotto in questi anni - una battaglia che è politica, giuridica e culturale - per spostare il baricentro del diritto penale non verso il *far west*, non verso violenze diffuse, ma verso la tutela del cittadino, del commerciante, della famiglia, affinché anche la magistratura faccia i suoi accertamenti, ma non ritenga di avere di fronte dei criminali, bensì delle vittime che non possono subire il supplizio di un altro processo.

poi, se altri sono collocati altrove, è problema loro. Il nostro è anche un voto a favore di uno dei cardini, dei temi principali del centrodestra: più sicurezza, più tutela per il cittadino, più legittima difesa. Con questa coscienza e con questa coerenza siamo lieti che questo provvedimento sia arrivato al suo passaggio finale: si poteva fare di più, prima e meglio, ma ci accontentiamo in attesa di archiviare un Governo che su altri versanti fa danni all'Italia. E siamo lieti di vedere almeno un pezzo del programma del centrodestra vincere con un voto che Forza Italia esprime con lo spirito di chi ha patrocinato queste tesi per primo, senza dover subire lezioni da nessuno, ma con quella coerenza che è la nostra

riguarda modifiche in materia di legittima difesa domiciliare ed eccessi colposi e interviene anche relativamente ad alcuni reati contro il patrimonio e sul delitto di violazione di domicilio. È vero che la materia è stata oggetto di modifiche con la legge n. 59 del 2006, che ha introdotto l'ipotesi della legittima difesa domiciliare, ma non è vero che quella riforma possa oggi considerarsi del tutto esaustiva. La legge non è statica e men che meno la dottrina e la giurisprudenza. Per affrontare le esigenze della società che cambia e si evolve continuamente, la legge deve allo stesso modo aggiornarsi sempre a tutela delle garanzie costituzionali nei confronti di ogni cittadino. È innegabile che oggi siano cambiate le condizioni sociali ed è fuor di dubbio che il legislatore non possa accontentarsi di aver riformato una legge nel passato, ma debba necessariamente intervenire per rendere i testi normativi adeguati ai tempi. L'istituto della legittima difesa è collocato normativamente tra le cause di giustificazione del reato e ha la sua ragion d'essere proprio nella necessità di autotutela della persona, quando non è possibile la tutela diretta da parte dell'ordinamento. - e lo dico ai colleghi della sinistra - è la stessa normativa che riconosce una speciale deroga, entro determinati limiti, alla prerogativa dello Stato dell'uso della forza. L'articolo 1, di modifica del secondo comma dell'articolo 52 del codice penale, introducendo l'avverbio «sempre» e così affermando che sussiste sempre il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa, trova finalmente una soluzione ai limiti della liceità della legittima difesa, che la presunzione legale introdotta nel 2006 non era riuscita a superare, eludendo di fatto il principio della presunzione assoluta. Con l'introduzione del quarto comma dell'articolo 52 del codice penale viene sancito il sacrosanto diritto all'autotutela, considerando sempre in stato di legittima difesa chi, di fronte agli atteggiamenti minacciosi posti in essere con l'uso di armi o altri mezzi di coercizione fisica, reagisca prontamente in difesa della propria vita o della propria o altrui incolumità. E questo non significa che non subirà un processo, perché l'azione penale in Italia è obbligatoria, proprio ai sensi della nostra Costituzione. Nel testo, poi, viene considerato il tema dell'abuso della scriminante integrativo alla legittima difesa. All'articolo 2, pur rimanendo identica la definizione che riconduce all'eccesso colposo, di cui all'articolo 55 del codice penale, vengono introdotti due commi, che escludono la responsabilità di chi abbia commesso il fatto in caso di minorata difesa o di grave turbamento, derivante proprio dalla situazione di pericolo. Inoltre, l'articolo 7 interviene anche sul piano civilistico della legittima difesa e dell'eccesso colposo, normando ulteriormente l'articolo 2044 del codice civile, con con la specifica che, nel caso di legittima difesa domiciliare, per cui è esclusa la responsabilità, *ex* articolo 52, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, è esclusa anche la responsabilità di chi ha commesso il fatto. Questa modifica è resa necessaria per impedire che l'autore del fatto, se assolto in sede penale, debba essere obbligato a risarcire il danno derivante dallo stesso evento in sede civile. Fino a oggi, le vittime, oltre a subire anni di processi, che le portano a rivivere quotidianamente le scene di violenza subite, quando ce la fanno, hanno dovuto risarcire con migliaia di euro ladri e aggressori, con gravi conseguenze, quindi, dal punto di vista non solo psicologico, ma anche economico, per se stesse e le proprie famiglie. Crediamo che queste norme abbiano, malgrado le discussioni strumentali di una politica di ristretti orizzonti, anche giuridici, un aspetto fortemente preventivo, in quanto soprattutto la disposizione dell'articolo 52 del codice penale, come modificata e combinata all'articolo 2044 del codice civile, agisce da deterrente, inducendo l'aggressore a desistere e a riflettere prima di porre in essere l'azione delittuosa, considerate la possibilità per la vittima, determinata ora dalla legge, di difendersi, se in determinate condizioni, e la negazione di qualsivoglia risarcimento monetario in sede civile, che spesso rende la vittima ulteriormente penalizzata. È proprio in quest'ottica, che molto spesso vede aggressori lautamente risarciti e beneficiati, in determinati casi, con la sospensione condizionale della pena, che si inserisce la subordinazione di tale concessione al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa, nei casi di condanna per furto in appartamento. Solo i miopi vedono il riferimento discriminante nell'unico elemento economico e non riescono a scorgere il lato preventivo della norma e l'azione di deterrenza a commettere il reato, considerato che queste azioni solitamente sono poste in essere da chi, non possedendo alcun capitale finanziario, va alla ricerca indebita di quello altrui. Altri elementi deterrenti della legge rientrano nell'inasprimento del quadro sanzionatorio per i reati di violazione di domicilio, furto in abitazione, furto con strappo e rapina, con previsione di ulteriore inasprimento delle pene per le ipotesi aggravate. Anche le disposizioni in materia di spese di giustizia, che estendono le norme sul gratuito patrocinio a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l'archiviazione o il proscioglimento e il non luogo a procedere, con decorrenza dell'onere dall'anno 2019, testimoniano la volontà di questa maggioranza di garantire e tutelare ogni cittadino che agisca nella legittimità della difesa. L'intervento legislativo in tema di legittima difesa ed eccesso colposo, nei termini in cui lo abbiamo concepito ed elaborato, si è reso necessario per porre fine ai casi di inciviltà che sempre più spesso costringono tutti noi a rinunciare alle nostre abitudini, alla nostra vita privata anche all'interno delle nostre abitazioni e delle nostre attività commerciali, professionali e imprenditoriali, per colpa di azioni criminose poste in essere da chi non ha il minimo senso civico di rispetto per l'altro. Non esistono giustificazioni per chi si introduce in un'abitazione privata, tanto più se la finalità è per delinquere, malmenare, violentare e spesso anche uccidere. E non hanno importanza i numeri o le statistiche relative ai procedimenti discussi o esistenti nei tribunali perché, se anche si trattasse di un solo caso, avremmo l'obbligo, con il potere legislativo a nostra disposizione, di intervenire in quanto garanti della legalità dello Stato. Fedeli a questo ruolo e ai princìpi di giustizia e legalità fondanti del MoVimento 5 Stelle e in cui ognuno di noi si riconosce, abbracciando simbolicamente tutti i familiari delle vittime e continuando a stare accanto a chi ce l'ha fatta, esprimiamo voto favorevole all'approvazione del provvedimento

tutto il Gruppo - sottolineo tutto il Gruppo - del Partito Democratico, dai membri del Gruppo Misto appartenenti a LeU, dalla senatrice Bonino e dal senatore dal senatore del Partito Socialista Nencini. Questa mozione chiedeva, Presidente, un chiarimento importante per quello che riguarda il patrocinio.

Mi risulta che siano vietate le foto in Aula, Presidente.

non nel nome dello Stato; un congresso dove parleranno persone che hanno solo l'interesse a discriminare tra famiglie di un certo tipo e altre di altro tipo. La cosa grave, signor Presidente, è che vi parteciperanno tre Ministri

perché alcuni Ministri, che amministrano e governano nel nome di tutti, nel rispetto della Costituzione, non possono prestarsi ad ambigue ambigue discussioni discriminatorie: la scuola è pubblica e resta tale. Il Ministro dell'interno faccia il Ministro dell'interno per tutti e per tutte le famiglie. Le famiglie sono tutte uguali: quelle di sposati, di uniti civilmente, le famiglie monoparentali, le famiglie monogenitoriali. Non è accettabile che, sotto lo scudo della Repubblica, si discrimini. *(Applausi

presentato un'interrogazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a proposito di un importante intervento di mitigazione acustica che deve essere realizzato dalla società Milano sul territorio del Comune di Buccinasco. Una serie di lungaggini burocratiche sta impedendo a quell'opera, finanziata da parte della concessionaria, di poter essere eseguita. L'interrogazione non è stata ancora evasa e, quindi, chiederei alla Presidenza di voler sollecitare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti affinché dia una risposta. A me non interessa tanto la risposta formale all'interrogazione che ho presentato quanto lo smuovere una penna dal banco del Ministero e del dirigente competente, il quale deve semplicemente approvare un piano finanziario che la società concessionaria ha presentato ormai da tempo, che è in ritardo e ancora non viene approvato dal Ministero. Solo con l'approvazione di quel piano finanziario l'opera di mitigazione acustica

Presidente, intervengo per richiamare le attenzioni del nostro ordinamento e, quindi, del Ministro competente su una questione autostradale che ha visto andare in onda qui anche un pezzo di spettacolo tra un interrogante civetta e il Ministro rispondente. Il decreto-legge per Genova ha assegnato 192 milioni di euro per lavori urgenti sull'autostrada A24-A25. seguito, abbiamo avuto la legge di conversione e per tre volte il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha sbagliato a redigere il decreto ministeriale, poiché è stato omesso il concerto dell'Ufficio centrale di bilancio dello stesso Ministero. La contabilità pubblica è costruita su una coppia di consistenze finanziarie, per cui ci sono la contabilità di cassa e quella di competenza: i 192 milioni di euro per gli interventi urgenti per la messa in sicurezza hanno avuto 162 milioni di euro in cassa e 30 milioni in competenza; nei fatti, da settembre, c'è una specie di pendolo di Foucault che non rende disponibili tali risorse. Intervengo quindi per richiamare le attenzioni dell'ordinamento e, attraverso di esso, del Ministro e del Ministero affinché si allineino linguaggi e documenti, per fare in modo che quelle risorse producano cantierizzazione tute di operai capaci di realizzare interventi. Ad oggi, quell'autostrada necessita di oltre 2 miliardi di euro di lavori: 192 milioni di euro sono in pancia al Ministero e circa 461 sono stati già utilizzati dal 2003 ad oggi.

Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per portare l'attenzione di quest'Assemblea su Cesare Battisti, terrorista più volte condannato, evaso nel 1981 dal carcere di Frosinone e per anni fuggitivo e latitante. Finalmente è tornato in Italia - in manette, se Dio vuole - grazie a un'operazione di polizia internazionale che l'ha condotto in arresto lo scorso 12 gennaio a Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia. Battisti è stato riconsegnato alle patrie galere e trasferito nel carcere di Oristano, dove finalmente potrà scontare l'ergastolo e non più circolare a piede libero, prendendo il sole sulle spiagge del Sud America e sorseggiando una Nei giorni scorsi, le cronache hanno riportato la notizia che Battisti ha ammesso - finalmente e per la prima volta, lo sottolineo - le proprie responsabilità per i crimini che gli sono stati imputati. Per la prima volta, dopo decenni, Battisti si è dichiarato colpevole - li ha ammessi, come riportano i verbali degli interrogatori - di quattro omicidi, fine a quattro vite innocenti per un'ideologia assassina e vigliacca. Leggo testualmente le parole del terrorista, perché così si chiama: «Sono stato sostenuto nella mia latitanza da partiti, gruppi di intellettuali, soprattutto nel mondo editoriale, come sostegno ideologico e logistico»; «(…) ero ritenuto un intellettuale, scrivevo libri, ero insomma una persona ideologicamente motivata». Nei suoi racconti si apprende di una vita normale, l'apertura di un ristorante, la scrittura di libri e la collaborazione con riviste, come nulla fosse, signor Presidente. Meno male che sono arrivati Bolsonaro in Brasile e Matteo Salvini in Italia, che finalmente hanno permesso di riportarlo nel nostro Paese e consegnarlo alla giustizia. Caro Presidente, mi avvio a concludere con una riflessione. L'ammissione degli omicidi da parte di Battisti non può che farci pensare a quegli intellettuali, scrittori, giornalisti, esponenti della sinistra *radical chic* che in tutto questo tempo si sono ostinati a difendere Cesare Battisti senza se e senza ma, come se fosse un perseguitato o la vittima di una persecuzione politica. E invece no, signor Presidente: era solo una persona che fuggiva dalle proprie responsabilità e dalla giustizia. Il problema di costoro è se il ministro Salvini indossi o no la giacca delle Forze dell'ordine e non se un assassino sia assicurato alla giustizia. Concludo con un invito a questa sinistra: continuate così;

fu protagonista, a livello locale e nazionale, di quella rivoluzione culturale, prima ancora che nella medicina e nella psichiatra, guidata dalle idee e dalle azioni di Franco Basaglia. Fu una rivoluzione certamente nel nostro Paese, ma, per il suo impatto, anche a livello internazionale. Ernesto Buondonno arrivò a Fermo, da giovane psichiatra, per lavorare nell'ospedale psichiatrico, quello che un tempo veniva chiamato manicomio. Negli anni Cinquanta, quando arrivò nel nostro Paese, la diagnosi della malattia mentale equivaleva a una vera e propria sentenza di morte e nei manicomi c'erano contenzione, isolamento e privazione

una malattia così angosciosa e dolorosa. Signor Presidente, il manicomio era l'emblema di una logica sociale volta anche all'annientamento del diverso. Ernesto Buondonno, con Franco Basaglia e tantissimi altri psichiatri, fu invece protagonista di un altro modello di psichiatria, quella che poi è stata chiamata psichiatria democratica, e delle lotte per trasformare i manicomi in comunità terapeutiche e, soprattutto, per superare i pregiudizi e lo stigma e abbattere i muri. Nel 1974 egli fu protagonista dell'apertura del manicomio, qualche anno prima della cosiddetta legge Basaglia, che nel 1978 sarà un passo enorme in avanti per il nostro Stato di diritto contro la segregazione e l'emarginazione sociale

quel rispetto e quei diritti di cui oggi ci fregiamo e per cui siamo conosciuti in tutto il mondo. *(Applausi *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei portare all'attenzione dell'Assemblea e anche del Governo, nella speranza possa rispondere alle interrogazioni depositate, notizie di pratiche illegali poste in atto da UBI Banca, i cui vertici sono a giudizio per gravissimi reati a seguito di circostanziate denunce inoltrate a partire dal 2012 da Adusbef e da un ex parlamentare, Presidente dei piccoli azionisti di UBI, Giorgio Jannone. Questo processo va avanti grazie alla costanza e alla tenacia di alcuni magistrati, come il pubblico ministero Fabio Pelosi, e dagli ufficiali della Guardia di finanza, tutti trasferiti perché non dovevano indagare su quel sepolcro imbiancato. Si tratta di fatti gravissimi che vengono censurati e oscurati nel cui processo, purtroppo, la Banca d'Italia neppure si è costituita parte civile. IWBank, l'istituto *online* del gruppo UBI, tra il 7 maggio 2008 e il 14 maggio 2014 avrebbe senza controlli antiriciclaggio per la notevole somma di 1.000 miliardi di euro - ripeto, 1.000 miliardi - senza le adeguate verifiche sulla titolarità effettiva delle somme movimentate su 104.000 dei 140.000 conti e con esami incompleti sugli altri 36.000. Il buco negli accertamenti obbligatori ha riguardato 49 milioni di operazioni su titoli e strumenti finanziari. Per quelle vicende, il pm di Milano Elio Ramondini lunedì scorso, 25 marzo, nel processo con rito abbreviato davanti al giudice per le udienze preliminari del tribunale Cristina Mannocci, ha chiesto la condanna a due anni e sei mesi per ciascuno dei 14 indagati nel procedimento in cui sono imputati anche in base alla legge n. 231 sulla responsabilità degli enti. Per questi gravissimi comportamenti, signor Presidente, ieri Bankitalia in tarda serata, solo dopo una decina di anni dall'inizio delle violazioni, ha diramato un comunicato in cui rende nota la decisione del direttorio dello scorso 8 marzo con cui è stata comminata al gruppo UBI la sanzione di 1,2 milioni per violazione delle normative antiriciclaggio. Sollecito quindi il Governo a rispondere sulla vicenda descritta e sulla direttiva europea sull'onorabilità dei banchieri, in applicazione della direttiva europea 2013/36 del 26 giugno 2013, che fa decadere dalla carica l'amministratore semplicemente indagato in vista dell'assemblea di UBI del 12 aprile (fra qualche giorno) i cui accordi prevedono il rinnovo di Victor Massiah alla carica di amministratore delegato e di Roberto Nicastro, ex presidente del fondo che con 3,6 miliardi salvò le quattro banche, regalando a UBI tre delle quattro banche. Un fatto molto importante riguarda Assogestioni, la società dei fondi che non ha presentato per protesta alcun candidato. Concludo, signor Presidente, auspicando interventi drastici a tutela del risparmio, ritenendo gravissimi questi comportamenti, come ad esempio il rinvio dell'udienza in prossimità della prescrizione per i reati di truffa ed altri gravissimi reati a carico dei banchieri di Arezzo, che hanno azzerato i risparmiatori di Banca Etruria, dove ci fu purtroppo il suicidio di Luigino D'Angelo. *(Applausi dal Gruppo M5S.